L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1427: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese». Nel corso della seduta del 26 marzo scorso la 1a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea. Domando all'estensore del parere, senatore Villone, se intende intervenire.

Ricordo anzitutto che noi, nell'esprimere questa valutazione, guardiamo soltanto al testo iniziale del decreto e non alle modifiche introdotte dalla Camera,

Ricordo anche che, quando parliamo della valutazione della necessità e dell'urgenza, non dobbiamo pensare - questo l'ho detto altre volte, ma è bene ripeterlo e lasciarlo agli atti

riferibili al precetto costituzionale, in quanto - come è oramai acquisito nella nostra prassi costituzionale, nell'esperienza pluridecennale possiamo avere una urgenza e una necessità che si collegano alle scelte di Governo, alle scelte di indirizzo politico: un obiettivo che il Governo assume come centrale, come necessario nei tempi più brevi ai fini della propria azione politico-amministrativa. Non dobbiamo nemmeno guardare, per l'urgenza e la necessità, a singole parti dell'atto normativo. È chiaro che, se esaminiamo qualunque decreto-legge, rigo per rigo o comma per comma, ne troveremo

Credo che queste condizioni vi siano nell'atto in discussione, né si può ritenere che vengano meno per le considerazioni che sono state fatte dai colleghi dell'opposizione e che sono state anche oggetto di dibattito pubblico, di interventi

attraverso una nuova e radicale disciplina per parrucchieri ed estetiste. Certamente, si può sorridere di questo. Io stesso, per la scarsità della materia prima che offrirei,

economico-produttivo, di eliminare vincoli e balzelli che molto spesso sono a carico dell'utente finale, del cittadino, e che certamente contribuiscono a rallentare l'azione delle nostre strutture economiche e produttive e delle nostre pubbliche amministrazioni, e contribuiscono quindi a volgere al basso la capacità competitiva del sistema Paese. Da questo punto di vista, come dicevo, superando le facili battute che non trovano spazio nella nostra discussione, abbiamo al nostro esame una serie di interventi normativi di un significativo rilievo.

da trattare in altra sede), il Governo si è riappropriato della questione e l'ha risolta. Se poi l'abbia risolta bene o male, è questione di merito che si valuterà nella discussione nella sede competente per materia. inoltre norme di trasparenza, che toccano questioni a tutti note, per esempio le tariffe aeree, che vengono ricondotte a verità. Noi tutti abbiamo sperimentato offerte strabilianti di voli ad un euro per andare da qui all'Antartide, che nascondono però una serie di costi occulti che il consumatore si trova ad affrontare. Ci sono norme rilevanti sulle assicurazioni, per eliminare i balzelli che vengono imposti all'assicurato per alcune operazioni del tutto normali nella gestione del rapporto contrattuale con la società assicuratrice.

Vi sono anche norme che riguardano punti nodali, per esempio la comunicazione unica. Il tema dello sportello unico, come tutti sappiamo, è stato ampiamente trattato e seguito

perseguito non solo attraverso questo decreto-legge, ma con una molteplicità di iniziative. Nell'ambito di tale dichiarata ed esplicita assunzione di un obiettivo fondamentale dell'azione di Governo, indubbiamente a questo decreto-legge

la disciplina dei decreti-legge è contenuta non soltanto nell'articolo 77 della Costituzione, ma anche nell'articolo 15 della legge

per venire incontro ad alcune incongruenze che la Corte costituzionale aveva posto in evidenza circa l'uso del decreto-legge.

Eliminiamo subito questo terzo parametro, perché il titolo del decreto-legge -

di fronte agli altri Paesi europei: qui si tratta di materie che nel titolo vengono completamente ignorate. Più particolari sono gli altri due parametri. Vediamo quello dell'omogeneità. come vi possa essere omogeneità se il provvedimento in discussione contiene norme in ordine ai seguenti temi, pur essenziali per la vita del Paese: tutela dei consumatori, mercato delle telecomunicazioni, informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete stradale e autostradale, trasparenza delle tariffe aeree, scadenza dei prodotti alimentari, servizi assicurativi, cancellazione di

L'eterogeneità è assoluta. E non si è fatto nemmeno lo sforzo di tentare di avere un'omogeneità delle materie indicate. Ci sono esempi eclatanti per quanto riguarda la seconda parte del decreto-legge,

mancanza di omogeneità, sicuramente si va incontro ad una disposizione che rende drammatica la scelta di trovare una scusa perché questo provvedimento possa essere urgente e necessario. Un altro parametro riguarda altro parametro riguarda le norme di non immediata applicazione in presenza di termini differiti.

Ne ha facoltà. MALAN *(FI)*. Signor Presidente, i requisiti prescritti dalla Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge sono la straordinaria necessità ed urgenza delle norme che si vogliono introdurre nell'ordinamento. In questo caso, non soltanto non sussistono in alcun modo tali requisiti in nessuno dei numerosi articoli e commi

dotate di maggiore contenuto e di meno apparenza, potrebbero essere positive, diventano confusionarie e generatrici di difficoltà di applicazione proprio per il fatto che, anziché essere introdotte attraverso

Di conseguenza, ci troviamo in una situazione in cui persino le norme che potrebbero essere positive diventano negative e quelle che intendono introdurre semplificazioni introducono complicazioni. Tali norme, proprio perché inserite da un giorno all'altro, anzi da un'ora all'altra, finiscono per generare contenzioso e complicare proprio laddove volevano semplificare. La mancanza di straordinaria necessità ed urgenza viene poi addirittura autodenunciata a chiare lettere nel provvedimento stesso, in particolare, ad esempio, nell'articolo 3, il cui comma 1

e, di conseguenza, di fare quanto in uno Stato di diritto la necessità della certezza del diritto dovrebbe imporre sempre. Invece no. Invece si vuole compiere una mossa pubblicitaria, un atto di immagine, facendo entrare in vigore tutto subito,

È stato approvato in Commissione alla Camera il 21 febbraio e l'esame in Aula alla Camera è iniziato il 9 marzo: sedici giorni che potevano essere utilmente impiegati per arrivare all'approvazione alla Camera e consentire al Senato di svolgere la funzione che la Costituzione gli assegna.

Presidente. Il meccanismo di questo decreto-legge è stato dettato da esigenze che nulla hanno a che fare con la buona legislazione. È stato dettato da ragioni di immagine, per la realizzazione di questa famosa lenzuolata che da varie settimane, prima ancora dell'emanazione del decreto-legge, veniva annunciata.

Per questo motivo abbiamo chiesto di portare in Aula il parere sui presupposti. Sul contenuto vi è molto da dire. Si tratta in gran parte proprio di quello che il provvedimento afferma di voler combattere: pubblicità ingannevole. L'abolizione dei costi di ricarica per i telefoni cellulari è semplicemente una questione di rimodulazione delle tariffe. Non vi sarà più il costo di ricarica, ma ci saranno altri costi, che verranno caricati su tutti gli utenti, anche quelli che prima, ad esempio, sfuggivano in parte ai costi di ricarica acquistando ricariche di importo maggiore. Un'altra pubblicità ingannevole è contenuta nell'articolo in cui si introduce la cosiddetta,

dell'operatività dell'impresa, ma unicamente della sua tassabilità. Questo è sicuramente l'obiettivo che il Governo persegue con coerenza. L'intero provvedimento presenta problemi notevoli. Ad esempio, va citato il fatto che l'articolo 9 introduce, naturalmente per decreto-legge, modifiche ad un decreto-legge di appena cinque mesi prima, il cosiddetto Bersani 1, segno, anche questo, di autodenuncia dell'inadeguatezza del sistema del decreto-legge per realizzare riforme di questa portata. Non parliamo, poi, della farraginosità dell'intera struttura del provvedimento. Leggendolo articolo per articolo, constatavo con piacere che gli articoli 6 e 12 erano stati soppressi. Certo, sono stati soppressi per poi essere introdotti nel grande guazzabuglio dell'ultimo articolo

che sottrae la facoltà legislativa alle Camere e in particolare al Senato. Tutte queste norme possono essere affrontate tranquillamente con il procedimento ordinario di formazione delle leggi, in cui tutti possono offrire il proprio contributo, maggioranza e opposizione;

siamo sconcertati per questo modo di agire del Governo che sembra interpretare, sempre più a modo proprio, addirittura anche la Costituzione.

però, nella storia dell'ordinamento italiano, i casi straordinari di necessità e urgenza sono sempre stati vagliati con un estremo rigore. Se andiamo a leggere i contenuti di questo provvedimento, si tratta di misure a favore dell'economia, della negoziazione, delle liberalizzazioni, della concorrenza, ma nessuno degli argomenti toccati può essere incasellato in un caso straordinario di necessità e di urgenza. Dopodiché, Presidente, ci si dovrebbe chiedere perché questi provvedimenti alla fine subiranno l'imposizione della fiducia. Innanzitutto, è stata già introdotta un'altra variante costituzionale, cioè la fiducia impropria; noi non la conoscevamo, ma sappiamo che esiste una Costituzione reale e poi una Costituzione materiale, fattuale.

A questo punto, cari parlamentari, riponete le vostre aspirazioni o velleità di modificarlo perché non è più possibile, dal momento che non ci sarebbe più tempo per riproporlo o riesaminarlo in seconda battuta. Ci si dovrebbe, a questo punto, interrogare; ci dovrebbe rispondere il Governo perché questo provvedimento, estremamente urgente al punto da non potere nemmeno quasi essere discusso, è stato fermato ben cinquantuno giorni alla Camera. Avrebbe dovuto essere stato

Non si possono pertanto non condividere le pregiudiziali di costituzionalità per questo disegno di legge di conversione; ma perché sulle riforme il Governo rinuncia addirittura al confronto parlamentare? Si tratta di questioncine, forse neanche tanto significative o importanti, che però innovano, modificano. Insomma, sarebbe come dire che solo il Governo sa interpretare i bisogni del Paese, tanto da non avere nemmeno bisogno del contributo delle Aule parlamentari. Era un po' come succedeva in quegli anni bui del Cristianesimo in cui si doveva convertire tutti, volenti o nolenti, a colpi di crocifisso; questo è ciò che sta facendo in questo momento il Governo nei confronti delle Aule parlamentari. Mi si scusi (magari poi si entrerà nel dettaglio), ma che urgenza sussiste di porre

della legge di conversione» - sta a significare che chi non li avesse nemmeno sa dove andare a recuperare tabelloni elettronici per esporre quelle informazioni che da domani saranno obbligatorie. Credo che nessun costruttore di queste apparecchiature sia in grado di fornire ciò che si chiede su tutta la rete stradale e autostradale italiana, a meno che non si sia già fatto un accordo sottobanco con la Cina, e noi sappiamo come riescono in quel Paese a soddisfare *just in time* qualsiasi tipo di ordinazione provenga dalle nostre parti.

meritevole della massima attenzione, perché tutti allo stesso tempo siamo anche consumatori, ma con lo stabilire, per esempio, che su qualsiasi tipo di contenitore dovrebbe risultare chiaramente leggibile la data di scadenza del prodotto non si dice

e quindi riconoscere la sussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì. I senatori contrari alla sussistenza di tali presupposti e requisiti dovranno votare no. I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

sulla situazione di Mario Scaramella, da 94 giorni agli arresti in carcere: un presunto innocente per la Costituzione

segnalazioni da lui fatte asseritamente per fatti riferitigli da Alexander Litvinenko un anno e due mesi prima che fosse arrestato; cioè, nell'autunno del 2005 Scaramella segnala che ci sono dei terroristi ucraini armati di granate e lanciagranate che vogliono attentare alla vita di alcune persone, tra cui il senatore Guzzanti. Per un anno la procura non agisce in nessun modo, né cerca di ascoltare Alexander Litvinenko. Solo dopo la morte per avvelenamento di Alexander Litvinenko la procura si muove e arresta

Mario Scaramella, che segnalando le notizie agli organi competenti ha consentito che queste persone fossero arrestate, è in carcere. Il ministro Mastella - al momento impegnato al telefono nelle scorse giornate ha, direi con grande sensibilità, chiesto al direttore del carcere di Regina Coeli, dove è detenuto lo stesso Mario Scaramella, notizie di un detenuto. Tale detenuto è Danilo Coppola, che pare abbia tentato il suicidio. È segno di grande sensibilità umana da parte del ministro Mastella aver chiesto queste informazioni, ma sarebbe sensibilità umana e istituzionale

un'inchiesta sulla Commissione parlamentare di inchiesta; un attacco all'autonomia del Parlamento, che giustamente non ha portato a nulla. Ma direi che una risposta a queste interrogazioni è doverosa.

al ministro Mastella. I colleghi hanno posto solleciti ad interrogazioni da loro presentate

riguardante il decreto sulle cosiddette liberalizzazioni,

con i requisiti propri della procedura d'urgenza, quindi con oltre 40 firme di senatori. Lei capirà perfettamente che se questa interrogazione non viene messa subito in discussione perde la sua ragione d'essere.